Comunico che, in data 29 novembre 2008, è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze*: «Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi

Capisco che c'è un motivo di cautela perché si vuole evitare che ci si approfitti surrettiziamente di questa opportunità per menare il can per l'aia. Ammetto anche che si possa discutere la liceità dell'intervento sull'ordine dei lavori perché, se è manifestamente estraneo agli argomenti,

secondo cui «I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione». Chiedo, dunque, che su questa decisione si ritorni e, se per caso si ritiene necessario

Insomma, insisto sulla validità della nostra posizione. il suo pensiero e il delibato (non mi permetterei di parlare di deliberato), cioè quanto concordato nella Conferenza dei Capigruppo, non vi sia una sostanziale differenza. Lei stesso ha giustamente richiamato le esigenze e il diritto di ogni singolo parlamentare di intervenire in ogni momento dei lavori dell'Assemblea allorquando si dovesse sentire tenuto a segnalare iniziative, osservazioni, dinamiche parlamentari attinenti ai lavori d'Aula in corso di svolgimento. Non vi è dubbio che il diritto del parlamentare è sacrosanto quando interviene - appunto - sui lavori in corso di svolgimento e questo

Abbiamo una costante prassi di questo tipo di interventi che, seppure richiamati all'ordine dei lavori, in effetti, hanno introdotto elementi di significatività tale da meritare l'ingresso nel dibattito d'Aula, pur non essendo riconducibili all'ordine dei lavori.

quella significatività, quella importanza e quella straordinarietà che consente la deroga all'intervento attraverso il richiamo all'ordine dei lavori possano essere ripetuti in maniera tale da rallentare e condizionare l'organizzazione dei lavori d'Aula.

in relazione alla segnalazione di anomalie o richieste che attengono all'andamento dei lavori d'Aula in corso di svolgimento o su richiami al Regolamento, né impedirà mai a ciascun senatore di intervenire per segnalare fatti straordinari che meritano la conoscenza da parte dell'Assemblea. Comunque le posso assicurare, senatore Pardi, che, alla fine del dibattito svoltosi in Conferenza dei Capigruppo, si è concordato, con la condivisione della Presidenza e di tutti i Capigruppo, di portare l'argomento in Giunta per il Regolamento, perché io riconosco che questo tema merita un approfondimento nella sede a ciò deputata. Quindi, le

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino a sabato 13 dicembre. A partire da oggi pomeriggio sarà discusso il decreto-legge recante misure per fronteggiare la crisi dei mercati finanziari internazionali, già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Sempre nel corso di questa settimana, a conclusione dell'esame del predetto decreto, sarà discussa la mozione Bianconi ed altri sulla prevenzione e cura dell'osteoporosi. Dopo l'illustrazione potranno intervenire i Gruppi per dieci minuti ciascuno. Altre mozioni sollecitate dai Gruppi - in particolare la mozione Rutelli sulla pirateria e D'Alia e connesse sull'integrazione scolastica dei minori stranieri - saranno calendarizzate a conclusione della sessione di bilancio. Tenuto conto dei limitati argomenti previsti dal calendario di questa settimana, le sedute di venerdì 5 dicembre non avranno luogo. Per quanto riguarda i disegni di legge finanziaria e di bilancio, resta confermato che la 5a Commissione permanente ne concluderà 1'esame entro sabato 6 dicembre e che gli emendamenti per l'Assemblea dovranno essere presentati entro le ore 10 di lunedì 8 dicembre. La discussione congiunta dei documenti di bilancio avrà inizio in Assemblea martedì 9 dicembre, alle ore 11, e proseguirà nel corso della prossima settimana per concludersi entro sabato 13 dicembre. I tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi per complessive 30 ore, escluse le dichiarazioni di voto finali. Il calendario della prossima settimana reca inoltre l'esame dei decreti-legge sul disagio abitativo e sull'emergenza rifiuti in Campania, già previsti dal precedente calendario per la settimana corrente e tuttora all'esame della Camera dei deputati. Tali provvedimenti, ove trasmessi in tempo utile dalla Camera dei deputati e se conclusi dalle Commissioni competenti, saranno discussi dopo il voto dei documenti di bilancio, eventualmente tra la votazione finale del disegno di legge finanziaria e la votazione del bilancio, utilizzando l'intervallo necessario alla predisposizione da parte del Governo della Nota di variazioni, nel caso di modifiche apportate al disegno di legge finanziaria. Diversamente, la trattazione dei due decreti-legge o il seguito della medesima avverrà nella settimana successiva. Infine, nel corso della odierna Conferenza dei Capigruppo il Ministro per ì rapporti con il Parlamento ha annunciato che il decreto-legge n. 185, recante norme in funzione anticrisi, già presentato al Senato sabato scorso, sarà trasferito alla Camera dei deputati per ragioni di equilibrio di carichi di lavoro tra i due rami del Parlamento. La Commissione straordinaria per i diritti umani è stata convocata per la propria costituzione giovedì 4 dicembre, alle ore 9. In occasione del 60° anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, in apertura della seduta antimeridiana di mercoledì 10 dicembre, sarà commemorata tale importante ricorrenza. Si procederà inoltre nei prossimi giorni alla costituzione della Commissione straordinaria per il controllo dei prezzi e del Comitato per gli italiani all'estero.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Atto Senato n. 1230 reca il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 155 del 2008. Nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, il disegno di legge in titolo ha assorbito il decreto-legge n. 157 del 2008 (recante ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio), di cui si è conseguentemente disposta l'abrogazione. L'Atto Senato n. 1230 deve essere approvato entro il prossimo 8 dicembre, a pena di decadenza del decreto. Entrando nel merito del provvedimento, esso autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad adottare, fino al 31 dicembre 2009, una serie di misure straordinarie eventualmente necessarie per fronteggiare l'attuale crisi finanziaria, al fine di garantire la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio. Da questo punto di vista, il decreto-legge in esame appare in linea con le conclusioni del Consiglio dei ministri economico-fmanziari dell'Unione europea tenutosi lo scorso 7 ottobre. L'articolo 1 interviene sulla disciplina della capitalizzazione delle banche italiane, autorizzando - fino al 31 dicembre 2009 - il Ministero dell'economia e delle finanze a sostenere finanziariamente gli istituti bancari che si trovino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. L'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze riguarda l'aumento di capitale sociale delle banche e può intervenire attraverso la sottoscrizione diretta di nuove azioni - emesse in occasione di aumenti di capitale - attraverso la quale il Ministero diviene socio della banca emittente la concessione di garanzie statali per la sottoscrizione di aumenti del capitale sociale da parte di altri soggetti. L'intervento del Ministero, nei termini sopra esposti, risulta subordinato alle seguenti condizioni: l'aumento del capitale sociale non deve risultare perfezionato alla data del 9 ottobre 2008, e ciò evidentemente per evitare il restauro di situazioni di dissesto o di disagio finanziario che si fossero verificate

è necessaria l'adozione di un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi. La stessa durata di medio termine ai fini del restauro sta a significare evidentemente che il nostro sistema bancario non ha patologie tali

Le operazioni di sottoscrizione degli aumenti di capitale o di prestazione di garanzie possono essere realizzate alle condizioni di mercato ed anche con riferimento ad aumenti di capitale di società capogruppo di gruppi bancari italiani. Altresì, esse devono essere attivate sulla base di un esame istruttorio condotto dalla Banca d'Italia, relativo, tra l'altro, all'adeguatezza del piano bancario di stabilizzazione e rafforzamento presentato per la delibera di aumento del capitale sociale. Banca d'Italia, auditi in Commissione, hanno più volte ribadito l'assoluta serenità per il sistema bancario italiano, che rispetto agli altri Paesi certamente si attesta come quello più attrezzato e più adeguato alla bisogna, considerata la stabilità di tutte le banche italiane. Nel corso dell'esame presso la Camera, si è precisato che le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito delle operazioni straordinarie di cui sopra, sono prive del diritto di voto, il che certamente sta a significare quanto l'intervento di questo provvedimento non sia per nulla invasivo e per nulla

di assemblea ordinaria e straordinaria, il che conferma la volontà del Governo di voler dare soltanto atto di sostegno e solidarietà, al sistema bancario certamente, ma per quella via ai depositanti, ai risparmiatori, ai cittadini italiani e non anche di voler entrare nel sistema bancario dal quale anni orsono siamo definitivamente usciti. Queste azioni saranno riscattabili da parte dell'emittente, subordinatamente ad una verifica della Banca d'Italia, volta ad attestare che l'operazione non pregiudichi le condizioni finanziarie e di solvibilità della banca, né del gruppo bancario di appartenenza. Ciò evidentemente sta a significare che il Governo, ove dovesse entrare ove dovesse entrare nel capitale, non ne uscirà se non dopo che si sarà reso conto che non è più necessario il sostegno finanziario da parte del pubblico. Pertutto il periodo in cui il Ministero dell'economia e delle finanze detiene le partecipazioni non è possibile apportare sostanziali variazioni al programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata, senza una preventiva approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ciò va nel rispetto dell'equilibrio del rapporto di libera concorrenza che, pur nell'esigenza di tutela occasionale del sistema creditizio, si appalesa necessario per non violare le norme che con tanta difficoltà nel tempo abbiamo voluto far nascere, ovvero di concorrenza adeguata all'interno del sistema bancario nell'interesse superiore della fede pubblica e dell'utenza. Quindi, per tutto il periodo in cui il Ministero dell'economia e delle finanze detiene queste partecipazioni non ci possono essere interventi straordinari di sostegno. Inoltre, non si applicano alle azioni detenute dal Governo le norme del Testo unico sugli intermediari finanziari. Qualora la banca interessata dall'intervento dello Stato sia di tipo cooperativo (banche popolari), non trovano applicazione le soglie massime di partecipazione al capitale sociale (il che evidentemente vanificherebbe, ove occorresse, la necessità dell'intervento dello Stato se trovasse applicazione quella norma di limitazione), né si fa venir meno il principio del voto capitario. Questa norma, determinata dalla volontà della Camera dei deputati e che il Senato certamente confermerà, sta a significare ancora una volta l'attenzione del Governo e del Parlamento a questo ambito del credito cooperativo, che oggi ascende ormai al 15 per cento del credito concesso al sistema produttivo italiano. L'individuazione delle risorse con cui finanziare le operazioni di sottoscrizione o garanzia degli aumenti di capitale delle banche è rimessa ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia, ma sentite le Commissioni parlamentari. In ciò, quindi, si vede la volontà determinata del Governo, ma anche il rispetto assoluto per il Parlamento per una materia così delicata. Tra le modalità di finanziamento specificatamente indicate, è inclusa l'emissione di titoli del debito pubblico. L'articolo 1-*bis* autorizza, sempre fino al 31 dicembre 2009 (permane quindi l'opinione che trattasi di intervento di breve periodo), il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva al 13 ottobre 2008. Siautorizza, inoltre, un meccanismo di operazioni di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari. Questo per tentare di eliminare dal mercato quell'infezione che si è verificata con i cosiddetti titoli atossici che, per fortuna, nel nostro Paese, per quanto hanno dichiarato l'ISVAP, la Banca d'Italia e la Consob, ascendono a percentuali veramente minime rispetto a tutti gli altri Paesi d'Europa e rispetto al resto del mondo. L'articolo 2 disciplina l'ipotesi di "grave crisi" di banche o di gruppi bancari, dovuta anche alla presenza di problemi di liquidità. L'articolo 3 reca una serie di deroghe alla normativa civilistica, per quanto attiene alle garanzie relative ai finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia, poiché anche le banche estere in Italia potrebbero traslare per osmosi i problemi e le tematiche negative che hanno contratto con infezioni manifestatesi in altri Paesi del resto del mondo. L'articolo 4, comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, integra la vigente disciplina italiana in tema di garanzia sui depositi, aggiungendo ai sistemi di natura privatistica già presenti nell'ordinamento la possibilità di rilascio, da parte del Ministero dell'economia, di una garanzia statale a favore dei depositanti, che può essere concessa fino a trentasei inserito dalla Camera dei deputati, è finalizzato a razionalizzare la disciplina della liquidità giacente all'interno del sistema bancario e finanziario sui conti e sui rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente. Il fondo al quale vengono acquisite acquisite tali somme sarà utilizzato per finalità molto provvide nell'interesse della fede pubblica e delle categorie meno abbienti (si pensi all'utilizzazione che se ne vuole fare per la *social card*). Infine, l'articolo 5 reca le disposizioni di attuazione delle norme del decreto-legge in esame, nonché la copertura finanziaria degli interventi di garanzia statale sui depositi e dei finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità. Sugli schemi di decreto si prevede l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo dire che il provvedimento in esame, trattato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, ha avuto l'attenta considerazione di tutti i colleghi, nessuno escluso, appartenenti ad ogni partizione partitica. Si è registrato tale e tanto senso di responsabilità che, pur in assenza di tempo sufficiente per poter delibare il contenuto dei vari emendamenti e dei vari ordini del giorno, si è ravvisata l'utilità di dare facoltà a chi vi sta parlando di rendere un parere favorevole, con il voto favorevole della maggioranza ma con l'astensione dell'opposizione, proprio per quel senso di responsabilità che evidentemente è nella *ratio* del provvedimento stesso. Si vuole riconoscere attenzione sì al sistema bancario, ma inteso come spina dorsale del sistema produttivo italiano

All'interno della Commissione è emersa chiara la preoccupazione che il sistema bancario non stesse rispondendo con la stessa moneta a favore del sistema produttivo, ma non perché non intende operare (perché è il suo mestiere), per un malinteso senso di preoccupazione e di inadeguatezza a rimborsare i capitali da parte del sistema produttivo. Ecco, la voce che oggi si leva dal Parlamento all'indirizzo del sistema bancario è la seguente: voi delle banche riservate al sistema produttivo un atto di fiducia e di coraggio. Non abbiate paura, così come non ne ha avuta il Governo nel momento in cui ha adottato questo provvedimento, che vi fornisce ogni tipo di paracadute. Guai se da parte vostra, banche, non ci fosse all'indirizzo del sistema produttivo la stessa fiducia che il Governo ha ritenuto di riporre in voi! Siamo fiduciosi che le banche, che oggi si rivelano essere tra le migliori del mondo e certamente tra le meno portatrici di patologie di tutto intero il sistema bancario e creditizio d'Europa e del mondo, sapranno rispondere a tale atto di fiducia.

Presidente, credo che il decreto-legge in discussione dia il segnale vero sul sistema delle relazioni economiche del nostro Paese, del sistema bancario e del Governo. La relazione del senatore Costa, puntuale in ogni suo aspetto, ha dato il segno dell'indirizzo governativo su una materia così complessa e difficile nel momento in cui il Parlamento italiano si appresta a varare un provvedimento che serve sì a salvaguardare

in particolare, vi è necessità di aiutare il sistema bancario; ma anche le banche devono fare il loro dovere nel contrasto all'usura, nella lotta al riciclaggio, ma soprattutto devono denunciare i mali del Mezzogiorno e dell'economia,

Quella banca serve soprattutto per colmare i vuoti che oggi esistono nel Mezzogiorno d'Italia, quella banca serve per dare di nuovo fiato e sviluppo all'economia meridionale. Per questo insistiamo nel dire che questo provvedimento va approvato senza

ha detto - e molto si trova negli atti che poi ha assunto - che la crisi di cui stiamo parlando è una crisi finanziaria che paradossalmente è troppo semplice definire così perché si tratta di una crisi globale di cui sono chiari gli effetti, ma meno chiare le cause. Credo che l'atto di cui si chiede l'approvazione contenga molti elementi che riflettono questi presupposti che si condividono, ma che non riflettono le conseguenze che da questi presupposti si dovrebbero trarre. Effettivamente siamo di fronte - e i numeri di questa crisi lo testimoniano ampiamente - alla più grande

e le decisioni che verranno assunte dai Governi in relazione a una crisi di questa natura sicuramente resteranno sui libri di testo, ma soprattutto resteranno come conseguenza sull'economia complessiva del nostro Paese e sulla capacità che avrà il nostro Paese di reggere a un'ondata di questa natura che ci trova più deboli rispetto ad altri Paesi per tante ragioni più volte ricordate. Il provvedimento che stiamo esaminando effettivamente applica un principio nuovo anche sotto questo profilo: applica una sorta di tutela mediante prevenzione, nella consapevolezza che la promessa di sicurezza in una fase di criticità di questa natura è di per sé un valore strutturale.

il decreto sono già oggi valutabili, perché sostanzialmente due erano le finalità che si leggono nel testo e che vengono poi sottolineate dalla relazione.

che gli strumenti hanno dovuto registrare - sono sostanzialmente basati su un assunto che, come ho detto prima, è ampiamente condivisibile: ci sono una necessità ed un'urgenza straordinarie di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori. Pertanto, lo Stato con questi provvedimenti ha concesso garanzie sulle passività del sistema bancario con la finalità conclamata di metterlo al riparo da onde eccezionali che arrivano dai mercati internazionali. Questa è la prima finalità. La seconda finalità, direttamente conseguente, è assicurare nel contempo che la maggior sicurezza delle banche ovviamente si rifletta positivamente sulle imprese assicurando una regolare prestazione di credito.

i tempi di conversione ci consentono di esaminare gli effetti e quindi l'efficacia stessa del provvedimento. A distanza di poco meno di due mesi possiamo dire che certamente non è stato centrato

230 miliardi quale *plafond* depositato dai grandi gruppi bancari europei presso le rispettive banche centrali - devo dire che era zero prima del *crac* della Lehman Brothers a fronte di un'offerta di liquidità che è stata aumentata, proprio perché i provvedimenti assunti dai vari Governi sono stati tesi ad immettere liquidità, a 323 miliardi. a 323 miliardi. Questo ci dice sostanzialmente che poco più di 90 miliardi sono confluiti nel circuito interbancario e che quindi la ricaduta sulle famiglie e sulle imprese è stata pari a zero. qualcosa di non previsto nei libri di testo, vale a dire che, mentre tradizionalmente l'immissione di liquidità porta ad un'immediata, non dico totale, ma pressoché totale, circolazione di liquidità, in questo caso si è verificato caso si è verificato un effetto non immaginato: è prevalsa la prudenza per cui il sistema bancario ha accantonato la maggiore liquidità e non se ne è avvalso per riversarla sul sistema delle imprese; l'ha depositata presso le banche centrali temendo

l'effetto fondamentalmente previsto da questa norma, vale a dire garantire la disponibilità di grandi risorse pubbliche perché il sistema del credito continuasse ad esercitare la propria funzione, ossia far avere risorse a famiglie ed imprese. Allora, se questo è un effetto non realizzato e prima ancora della conversione del decreto in legge possiamo già constatarlo, ci si sarebbe aspettati evidentemente dagli

capire quali sono gli atti che occorre porre in essere perché l'effetto indicato e non ottenuto con questo decreto, il n. 155, possa essere effettivamente ottenuto ottenuto con atti successivi, non più con questo che è destinato ad essere approvato, a questo punto, così com'è perché ci troviamo in una situazione del tutto particolare e sostanzialmente parliamo di un provvedimento provvedimento vecchio, un provvedimento che possiamo archiviare, che ha avuto sicuramente un effetto positivo perché ha rappresentato un ombrello di rassicurazione emotiva (elemento immateriale che nelle crisi economiche ha una proprio validità), rispetto all'obiettivo finale dobbiamo effettivamente denunciare una carenza che non vediamo colmata con atti successivi. Il collega che mi ha preceduto ha sottolineato un appello al sistema del credito perché corrisponda in termini positivi alla disponibilità che il Governo e il Parlamento hanno dimostrato nel mettere a disposizione un grande paracadute. Io credo che non sia questo l'approccio giusto, nel senso che il rapporto con un sistema imprenditoriale quale quello del credito non è un rapporto a cui si chiede la gentilezza di corrispondere ad una nostra cortesia. Non è stata una cortesia quella istituzionale: è stata una scelta politica e tecnica molto chiara e molto precisa, a cui devono corrispondere comportamenti non lasciati alla cortesia di un sistema, ma normati attraverso disposizioni molto precise che tendano ad evitare che grandi risorse messe a disposizione servano a risolvere problemi aziendali e non problemi collettivi; le risorse collettive, infatti, servono a questo. Altrimenti, ci troveremo nella fastidiosa situazione, che in un momento di crisi va assolutamente evitata, di avere qualcuno che rompe e qualcun'altro che paga.

le proposte dell'Esecutivo che siamo chiamati ad approvare richiederebbero un'attenta analisi del momento di particolare crisi economica nazionale e mondiale che stiamo vivendo,

ha di nuovo rivisto al ribasso le attese già negative per il 2009. La crescita del prodotto interno lordo mondiale è ora prevista al 2,2 per cento (sono dati che ho desunto dal centro studi Banca Akros)

Siamo praticamente al di sotto del tasso di crescita della popolazione del pianeta, con un conseguente, reale, impoverimento globale. Nel complesso delle economie avanzate, si prevede una contrazione del PIL (meno 0,3 per cento) per la prima volta dalla seconda guerra mondiale, mentre per i Paesi in via di sviluppo la crescita,

il risultato dovrebbe essere decisamente più brutto in questo quarto trimestre, quindi è attesa una diminuzione nell'ordine di tre-quattro punti percentuali su base annua, che ne farebbe il peggior trimestre dal 1982.

ottimisti, perché sicuramente le misure che stiamo per mettere in campo insieme a tutti gli altri provvedimenti tampone aiuteranno il nostro Paese e quanto stanno facendo gli altri Paesi del nostro continente farà il resto. In Europa la discesa del PIL è causata soprattutto dall'estrema debolezza di Germania e Italia, è inutile nascondercelo. Il dato italiano

L'Italia torna in recessione, con un quadro che però questa volta ricorda molto il periodo 1992-1993, quando c'era la "liretta" e si poteva venire incontro a questi problemi causando tutti i guai che stiamo vivendo adesso. Non aggiungo altro, perché non voglio peggiorare il vostro pensiero sul futuro, a cui tengo moltissimo, e non intendo rivolgermi al passato che, però, pesa. Sappiamo che in questi giorni le autorità statunitensi lavorano su vari fronti per cercare di scongelare i mercati creditizi. monetaria che il Governo federale USA ha messo a disposizione del sistema del credito ammonta a ulteriori 350 miliardi di dollari. È interessante notare che il Tesoro USA, in pratica, riconosce che il problema principale è la patrimonializzazione degli operatori finanziari, ma anche che i fondi messi a disposizione devono essere utilizzati in diversi modi per massimizzarne l'efficacia. Nemmeno il collasso dei prezzi delle materie prime, che sta generando una precipitosa discesa dell'inflazione e quindi

È infatti atteso un forte aumento del tasso di risparmio, che nel quarto trimestre dovrebbe superare il 3 per cento (dall'1,3 per cento del terzo trimestre) che non genera alcuna ricchezza. Ecco quindi la necessità di un quadro di interventi articolato, di cui il tassello relativo al sistema finanziario è dato dall'atto Il Governo, con i decreti-legge nn. 155 e 157, ora unificati, non ha inteso prevedere un indiscriminato - come ho sentito dire - apporto finanziario alle banche. Ha piuttosto scelto la strada per generare nel sistema bancario una nuova fiducia tra gli operatori, anche se il sistema italiano non è stato particolarmente esposto alle sofferenze. Finora almeno è stato così e ci auguriamo che si possa continuare a dire così. Siamo in presenza di un provvedimento che non contiene la tecnica dello "*stop and go*" di qualche decennio fa, volta ad evitare la stagnazione e l'inflazione - come qualcuno

anche perché individua strumenti molto significativi di sostegno al sistema bancario, quali la ricapitalizzazione e lo *swap* di titoli, che prefigurano nuove forme di intervento pubblico nell'economia. Qualcuno ha avanzato che sia in atto una lotta di potere con il sistema bancario, ma questi provvedimenti non hanno natura coercitiva. Essi costituiscono strumenti di sostegno che le banche, se lo vorranno, potranno utilizzare senza che ciò incida sulla gestione delle banche stesse. Non per nulla i deputati hanno inserito, all'articolo 1, comma 3, lettera *a**)*, un emendamento per cui le azioni privilegiate, acquisite eventualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, per la ricapitalizzazione delle banche, saranno senza diritto di voto. Appare evidente l'intenzione del Governo di evitare un'impropria "statalizzazione" del sistema bancario, ma anche di scongiurare ogni riduzione della disponibilità di credito da parte delle famiglie e delle imprese. Gli interventi che dobbiamo approvare sono perciò mirati e molto circoscritti. Mi riferisco alla garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità. penso alle misure per sostenere il capitale delle imprese bancarie in difficoltà; oppure a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, modificato dalla Camera, in tema di garanzia sui depositi, laddove si aggiunge, ai sistemi cautelari di natura privatistica, una garanzia statale a favore dei depositanti. Il tassello che discutiamo è parte di una volontà del Governo molto chiara, Chi pensava che l'azione del Governo fosse circoscritta al sistema del credito si sbagliava. Non solo i risparmiatori saranno tutelati, ma milioni di famiglie potranno ricevere sostegno e migliaia di imprese trovare occasione di nuovo sviluppo. La crisi mondiale ha bisogno di una regia mondiale per limitare le ricadute sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese. Oggi questa regia appare più evidente e di questo l'Italia e il Governo Berlusconi recano una consistente parte di merito per quanto fatto sia in sede di Unione europea, sia nell'ambito dell'incontro dei venti Paesi più industrializzati del mondo. Anche il continuo richiamo del Presidente del Consiglio alla solidità del sistema economico italiano è parte di questa manovra. Tutti dovremmo sentirci coinvolti nel richiamare alla fiducia le famiglie e le imprese: essa è la base della ripresa e lo dobbiamo fare tutti. Ha ragione il Governo a voler rispettare, anche in questo momento difficile, l'impegno del contenimento del debito pubblico nel limite che ci eravamo prefissato: ciò sarà positivo per tutti e non ci sarebbe futuro se sin d'ora si cominciasse a dire che non manterremo gli impegni di Maastricht o se magari pensassimo a stampar moneta (io lo farei, ma non si può fare in quanto l'Italia ha una credibilità e questo Governo anche). Credo che ci attenda una crisi non breve. Se sarà così, sarà richiesta una compattezza nuova delle forze politiche; una compattezza che al momento non vedo perché mi pare ci sia ancora troppa ideologia in circolo. Penso che la prima regola per aiutare chi ha bisogno sia quella di avere i mezzi per farlo: non si distribuisce ricchezza

qualcuno dirà che le imprese vogliono socializzare le perdite. La verità è che ci siamo trovati di fronte ad un sistema finanziario che ha perso pezzi perché ha fatto ciò che non doveva e ha trascinato con sé chi lavora e chi produce davvero. A questo settore, all'economia finanziaria globale, sarà necessario rimettere regole chiare,

Presidente, se la situazione nazionale e internazionale è grave, nel Meridione è gravissima.

penso di dovermi occupare maggiormente, la fine del Banco di Sicilia o della Cassa di risparmio non è stata solo la ridisegnazione della storia del credito siciliano, ma anche quella di un progetto politico, sociale ed economico. Se da un lato, infatti, questi istituti avevano accompagnato i gracili processi di crescita di un secolo di economia isolana, dall'altro attorno ad essi si era definito un reticolo di micro e macro interessi, sia economici che politico‑sociali. Lo *shock* creditizio che si determinò con la fagocitazione di questi due emblemi della Sicilia rese ovviamente più semplice la ridefinizione complessiva del settore e, dopo tutto, meno conflittuale l'assorbimento di un lungo elenco di istituti di minore

nella debolezza della loro struttura patrimoniale e nella grave situazione della voce sofferenza, così come nella più complessiva fragilità competitiva nell'ambito di un settore, come quello creditizio, che si confrontava in quegli anni con l'aggressività della competizione globale, ma che, al contempo, serviva a definire un complessivo disegno di subalternità del sistema Mezzogiorno. Infatti sembrava inaccettabile, ai poteri forti del Paese, che il Sud, da un lato, lucrasse ampi flussi di spesa pubblica e, dall'altro lato, utilizzasse nello stesso Mezzogiorno il risparmio generato dalle famiglie mantenute dalla stessa spesa pubblica. Al sistema produttivo settentrionale non bastava più, in periodi di restrizione della spesa pubblica, che le famiglie meridionali utilizzassero in consumi di beni provenienti dal Nord buona parte del loro reddito. Era necessario ricanalizzare verso il Settentrione anche i risparmi. Dopo tutto, la loro idea era quella che i redditi meridionali trovavano la loro fonte nella richiesta nazionale ritrasferita al Sud mediante la spesa pubblica. Così, dovendosi riappropriare dei risparmi, lo strumento fu trovato nell'assorbimento dell'intero, o quasi, sistema creditizio. La Banca d'Italia iniziò a spulciare esageratamente i conti di banche e banchette e trovò, inevitabilmente, debolezze gestionali che giustificavano l'assorbimento da parte di istituti più grandi e moderni

sul piano del credito si trasformò in un processo inevitabile di modernizzazione che coinvolgeva, da Roma in giù, istituti come il Banco di Roma, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e l'intero sistema delle Casse di risparmio meridionali. Ad essere travolte, nel silenzio generale, fu anche un enorme reticolo di banche, di piccole o piccolissime dimensioni, che non appartenevano alla storia d'Italia, a quella più modesta di tanti territori dei quali avevano tracciato un percorso di sviluppo locale. Gli effetti sono noti: una miriade di piccole e piccolissime aziende e una moltitudine di imprese agricole o artigianali si trovarono, dall'oggi al domani, a dover contrattare la loro sopravvivenza con funzionari incapaci o impossibilitati ad analizzare i loro bisogni e con canali di credito sempre più asfittici. Era inevitabile. Il risparmio doveva finanziare nel Mezzogiorno solo debitori affidabili. Gli sportelli dovevano servire a rastrellare il risparmio più che considerarlo verso impieghi modesti come modesta è l'economia siciliana. A svilupparsi, piuttosto, era un sistema di captazione capillare del risparmio attraverso due strumenti: per i risparmi di dimensione più elevata erano disponibili tutti quegli strumenti di finanza creativa che si annidavano dietro il cosiddetto risparmio gestito, del quale gli istituti meridionali erano, e sono, intermediari; per rastrellare scientificamente i risparmi della povera gente ci si è serviti di tutti quei piccolissimi istituti di credito al consumo che stimolano e finanziano l'acquisto rateale di prodotti generati dall'apparato produttivo al di fuori del Mezzogiorno. Per le imprese siciliane restano o l'autofinanziamento o una concorrenza micidiale su un mercato del credito poco comprensivo delle nostre secolari difficoltà. È tutto perduto? In verità, come avviene in silenzio nel sottobosco dopo un incendio, la vita lentamente si riorganizza. In fin dei conti, in un mondo che si era strutturato su nuove ed ipertrofiche oltre che ipermoderne istituzioni (come le *investment banks*, che rastrellano risparmi senza fare banca), anche gli istituti tradizionali si sono salvati, pur se a stento, solo, appunto, facendo banca. Così i bisogni reali del micro-territorio vanno incontro ad una riorganizzazione, attraverso la silente crescita di un reticolo di nuove realtà, quali le banche di credito cooperativo che svolgono, senza enfasi, il ruolo di banche *retail* acquisendo risparmio ed erogando il credito a sostegno di una clientela radicata nel territorio in termini produttivi. C'è da esserne soddisfatti, ma contemporaneamente non possono essere enfatizzati esiti che si confrontano con una realtà debolissima sul piano produttivo e con fonti di risparmio in via di essiccazione ed esaurimento, tenuto conto del crollo del reddito del cosiddetto ceto medio. Questi micro-istituti, certamente benemeriti, se da una parte rassicurano una clientela mortificata dai comportamenti distratti e disattenti delle grandi istituzioni bancarie, dall'altra sopravvivono in una nicchia operativa dai margini risicati, potendo erogare prettamente credito di gestione, ma essendo fuori dal credito per investimento. In definitiva, l'abbandono da parte degli istituti nazionali del micro-credito ha aperto molti piccoli canali operativi a queste altrettanto piccole realtà creditizie. Ciò aiuta e può aiutare la sopravvivenza delle piccole attività produttive che costituiscono il tessuto della nostra economia. Sarebbe, però, impensabile poter costruire su queste realtà ipotesi di crescita, poiché questi istituti non hanno le risorse per assolvere tale ruolo: infatti, se solo deviassero dai loro comportamenti di buoni padri di famiglia finirebbero con il deragliare dai loro percorsi virtuosi. Promuoviamone dunque la nascita e guardiamo con affetto alla loro azione, ma comprendiamone anche i loro limiti. Essi sono il sostegno di un'economia di pura sopravvivenza che necessita di credito e di pure operazioni gestionali di breve periodo, ma contemporaneamente sono istituti impossibilitati a finanziare progetti di crescita di lungo termine.

Infine, la loro funzione va collocata entro aree che non godono di redditi inesistenti, ma di aspettative positive, almeno nel breve periodo. La loro clientela, dunque, sia sul piano dei depositi che degli impieghi si appalesa come riferimento fragile ed il rapporto complessivo si attesta più su vincoli fiduciari che su aspettative di ampi grado, tuttavia, di contrastare almeno nell'attuale contesto economico regionale, nazionale ed internazionale la rapace attività dei grandi istituti bancari. Questi ultimi, peraltro, iniziano ad avvertire il peso della loro disattenzione nei confronti del territorio. Non è un caso, infatti, che Unicredit abbia riproposto di recente la presenza del logo «Banco di Sicilia» nel tentativo di riposizionarsi attraverso una identità sul mercato del credito. C'è da augurarsi che non si tratti soltanto di una penosa attività di *marketing*.

il disegno di legge in discussione predispone uno schema di intervento a sostegno degli istituti di credito in crisi. Al momento è solo un'ipotesi di intervento, un'arma carica che non ha ancora sparato alcun colpo e che speriamo resti nel cassetto e sotto chiave. In ogni caso, non possiamo escludere l'impiego di risorse pubbliche per sostenere le banche in difficoltà attraverso l'acquisto di azioni privilegiate o altre forme di intervento pubblico. L'ultima volta che un Ministro ha ritenuto giusto lasciar fallire una banca è stato il 14 settembre 2008, quando Henry Paulson ha spiegato ai manager della Lehman Brothers che se la sarebbero dovuta cavare da soli. Ebbene, quei manager hanno dichiarato fallimento ed hanno trascinato con loro imprese e risparmiatori di tutto il mondo, diffondendo il panico sui mercati. A causa di quel panico oggi migliaia di padri e di madri hanno perso il lavoro ed altri lo perderanno nei prossimi mesi. Sarebbe il momento di chiedere conto degli anni di *rally* in Borsa, delle *stock option* e dei vari *bonus* milionari a favore dei manager. Oggi possiamo dirlo: incompetenti; arroganti ed incompetenti. Invece l'Italia e tutte le principali economie sviluppate hanno approvato norme d'emergenza per garantire la sopravvivenza di quelle stesse banche. È la cosa più ingiusta da fare e al tempo stesso l'unica possibile per evitare ulteriori danni. Gli economisti hanno un termine tecnico per descrivere questa situazione: azzardo morale. Non credo sarei in grado di spiegarlo alle madri e ai padri che hanno perso il lavoro in questi mesi. Quello che si discute in Aula non serve solo a salvare le banche ma anche ad evitare che le imprese, specialmente quelle di dimensioni ridotte, smettano di ricevere i finanziamenti, rimandando gli investimenti e licenziando personale. Per questo l'efficacia della norma dipenderà dai programmi di stabilizzazione e rafforzamento delle banche e dalle loro politiche di credito. Dipenderà da quanto contenuto in quei documenti se l'intervento che approviamo oggi sarà un favore alle banche che hanno causato la crisi, o alle famiglie che questa crisi l'hanno subita. Mi auguro che vengano tenute sotto controllo la politica dei dividendi delle banche e la remunerazione dei manager. E visto che ci apprestiamo a destinare fondi pubblici a favore degli istituti di credito sarà necessario avere qualcosa in cambio nell'immediato, a favore dei clienti, come politiche più amichevoli per i mutui o finanziamenti agevolati agli artigiani e alle piccole imprese. Possiamo anche chiedere un ulteriore sacrificio al contribuente, ma dobbiamo portare a casa qualche risultato perché i nostri mutui costano lo 0,5 in più rispetto a quelli degli altri paesi europei. E perché le principali banche del Paese stanziano un miliardo e mezzo di euro a favore di un singolo speculatore finanziario sull'orlo del fallimento e e chiedono il rientro dai fidi a migliaia e migliaia di piccoli imprenditori? Attenzione! Le banche italiane non sono In questi anni hanno fatto importanti acquisizioni all'estero ed hanno sostenuto imprese come Alitalia - e qui un po' tra virgolette - o la FIAT che da sole sarebbero scomparse, lasciando a casa centinaia di migliaia di lavoratori. Eppure oggi hanno fallito nella loro principale missione: la gestione del rischio. Non si sono dimostrate in grado di mettere il proprio patrimonio al riparo da avventurose speculazioni. Per questo serve una nuova stringente regolamentazione, il più possibile uniforme in tutti i sistemi europei. E poi una riforma specifica per gli istituti di credito italiani, che elimini quei conflitti di interesse che hanno generato i casi Parmalat e Cirio. Oggi vi è un tornado e dobbiamo sbarrare le finestre e rinforzare i tetti. Domani dovremo rifare daccapo le fondamenta, riscrivere le regole del gioco. è la possibilità che lo Stato guadagni da un intervento nel capitale delle banche: acquistare oggi che le quotazioni sono molto basse e rivendere a crisi finita quando i listini saranno tornati ai livelli ragionevoli. Può essere addirittura un affare! In ogni caso non credo che il compito del Governo sia fare *trading* o speculare sui titoli. Mi accontenterei di non mettere in pericolo il bilancio. Proprio questo è il punto. Le garanzie offerte dal Tesoro hanno un senso solo se lo stesso Tesoro non ha difficoltà di finanziamento sul mercato. Non vi sono segnali in questa direzione. Ciò non toglie che un debito pubblico ben al di sopra del 100 per cento del PIL non consenta spese fuori controllo. Non possiamo stanziare altre decine di miliardi a pioggia, come sento chiedere dall'opposizione, e non possiamo neanche permetterci uno sciopero generale. Non è nelle nostre possibilità; non oggi, non con questa crisi in corso. Per questo faccio un appello alle opposizioni e alla CGIL: fermatevi. Fermate lo sciopero. Ovviamente lo sciopero è un diritto sacrosanto, sancito dalla nostra Costituzione, ma per il bene dell'Italia oggi fermatevi. Non è il momento di dare segnali negativi ai mercati: già dubitano della solidità delle nostre banche, non facciamoli dubitare della capacità di uno Stato di tenere sotto controllo la spesa e il debito pubblico.

di fronte ad una delle più gravi crisi finanziarie che ha sconvolto gli assetti portanti e le regole di un capitalismo senz'anima e senza alcuna etica, basato principalmente sulla rincorsa forsennata all'indebitamento (cioè quella creazione del denaro dal nulla della dottrina Bush-Greenspan-Paulson), di fronte ad una crisi annunciata almeno un lustro fa da alcune inascoltate cassandre, che sta mangiando l'economia reale ed il futuro di giovani generazioni destinate al precariato perenne, l'Italia dei Valori aveva offerto disponibilità per cercare soluzioni idonee ad attenuarne gli effetti. Ma per quanto ci siamo sforzati, per quanto anche oggi in Commissione finanze abbiamo cercato di trovare delle convergenze, da parte della maggioranza, che va avanti a colpi di fiducia e che, a differenza di tutti gli altri Governi - dall'America alla Francia, dall'Inghilterra alla Germania - ritiene nella sua assoluta autosufficienza di risolvere le questioni di politica economica con le carte di carità da 40 euro al mese salvo poi chiedere a cose fatte collaborazioni, non abbiamo trovato alcuna sensibilità ad accogliere le proposte dell'opposizione democratica, salvo qualche sparuto ordine del giorno. cosiddetto decreto salva banche del Governo, invece di andare verso la giusta direzione nell'individuare gli autori del disastro finanziario, che, seppur in maniera meno grave, ha ugualmente colpito il sistema bancario (chi afferma il contrario vada a leggersi le quotazioni e le perdite in Borsa degli ultimi tre mesi), rappresenta una misura premiale a favore di banchieri che hanno frodato almeno un milione di risparmiatori negli ultimi cinque anni, appioppando loro *bond* bidone, da Parmalat a Cirio, dalle obbligazioni argentine alle polizze tossiche Lehman. pone la finalità di ricostruire una fiducia tradita, auspicando anche che i consumatori delle piccole e medie imprese, strozzate dalla stretta creditizia, possano fidarsi di quelle stesse banche che non si fidano tra loro, come dimostra la crescita dei depositi presso la Banca centrale europea, che a settembre era pari a 48 miliardi di euro e, un mese dopo, a 280 miliardi di euro. La BCE pompa liquidità che, invece di essere utilizzata per finalità produttive,

su un conto presso la stessa Banca centrale europea, ad un tasso di interesse inferiore dell'1,5 per cento rispetto a quanto pagato dal mercato interbancario. I banchieri qui non si prestano soldi fra loro, non finanziano le imprese, specie le piccole e le medie, alle quali vengono anche richiesti rientri degli affidamenti con un preavviso di ventiquattro ore. Chi parla di un sistema bancario sano (oggi ho ascoltato anche l'ex governatore della Banca d'Italia Fazio, che è salito in cattedra) vada a vedere gli andamenti dei listini di ieri, dove non solo le *big* del settore, come Unicredit e Intesa, hanno registrato ulteriori ribassi, ma anche il Banco Popolare ha subito un crollo del 16,36 (stamattina perdeva un ulteriore 14 per cento, quotando poco più di 5 euro), trascinato dal fallimento della trattativa di Banca Italease (ce la ricordiamo) con i tedeschi di Dz Bank, che ha perso a sua volta il 14 per cento scendendo al minimo assoluto di 2,71 euro. Tutto ciò senza che questi signori banchieri, novelli padroni del vapore che il Governo si ostina a voler salvare, sentano il dovere, non dico di ricorrere alla virtù rara dell'istituto delle dimissioni o di restituire premi e prebende che si sono elargiti a piene mani, ma almeno di fare un minimo di autocritica; neppure quello. Il decreto salvabanche, mentre garantisce agli istituti di credito finanziamenti indefiniti, perciò illimitati (una vera e propria fideiussione *omnibus*, trasformando tali linee di credito in *bond* perpetui per far fronte alla crisi patrimoniale e di liquidità di alcuni istituti di credito) non offre alcuna tangibile garanzia alle piccole e medie imprese alle quali le banche stanno inviando lettere di rientro. Ho molte lettere di rientro

da garantire attraverso un fido. La banca in questione è Unicredit, che - come tutti sappiamo - è stata indicata come tra le prime banche da soccorrere. Con questo decreto il Governo diventa complice delle malefatte di un sistema bancario che utilizza le norme secondo le proprie convenienze, come la simmetria dei tassi d'interesse, il ricorso normale all'anatocismo, il rimborso alla francese dei prestiti nell'ammortamento dei mutui usurari (prima gli interessi poi il capitale), la violazione della surroga e della portabilità dei mutui, ma soprattutto di quello che è stato definito il sistema Zaleski, ossia un fiduciario delle banche, a cui è stata erogata

hanno poi messo a garanzia come pegno di quei crediti allegramente elargiti. Non voglio usare, signora Presidente, onorevoli colleghi, termini forti anche se la tentazione sarebbe quella di utilizzarli; utilizzarli; però siamo nell'Aula del Senato per cui devo trattenere l'indignazione rispetto a questo sistema bancario che oggi si dice - è riuscito a ristrutturare i debiti della Tassara con la banca presieduta - ricordiamolo - dal professor Bazoli,

Il decreto salvabanche non risolve neppure il grave conflitto di interessi di banche, che invece di vendere agli sportelli prodotti finanziari più consoni al profilo di rischio dei clienti, che vogliono solo salvaguardare il frutto del loro risparmio ed avere la certezza di quotazioni trasparenti in caso di vendita anticipata e prima delle scadenze, promuovono e piazzano anche in questi giorni di tempesta finanziaria loro obbligazioni (invece dei richiesti titoli di Stato), che peraltro non hanno alcuna garanzia di trasparenza nelle quotazioni e che possono essere manovrate dalle stesse banche emittenti, con grave pregiudizio e grave danno alla generalità degli utenti. Mi rendo conto che ci sono obbligazioni bancarie che sono 2,7 volte il patrimonio delle banche

come i metodi a volte illeciti di piazzare loro obbligazioni mediante un sistema premiante e con degli incentivi: montagne di *bond* che i risparmiatori dovranno rifinanziare, equivalenti a circa le metà del debito pubblico, ossia 34.200 euro in media di *bond* bancari per ogni famiglia. il Governo non ha voluto inserire alcuna norma per contrastare un malcostume noto, che portò a regalare una Ferrari Testarossa dall'ex amministratore della Banca Popolare di Lodi, Giampiero Fiorani, a quel dipendente che riusciva a piazzare più titoli avariati.

mentre i consumatori e le piccole e medie imprese, strozzate dall'avidità degli stessi banchieri, non hanno avuto alcuna misura tangibile per sostenere le loro attività. *(Applausi del

la crisi finanziaria globale ha colpito duramente il nostro Paese, l'Unione europea e un po' tutto il mondo. La stretta creditizia, la diminuzione dei prezzi delle abitazioni, il crollo delle Borse hanno effetti sempre più negativi sulla fiducia dei consumatori, sul consumo e sugli investimenti. La pressione sulle famiglie è reale. I portafogli di ordine delle ditte sono assai sguarniti. I settori che dipendono dal credito al consumo, come l'edilizia privata e l'industria automobilistica, hanno visto i rispettivi mercati subire un forte deterioramento in molti Stati membri. in discussione, varato in un momento di grande difficoltà e di grande panico, possiamo usare questo termine, forse sottostimando il momento che vivevamo a settembre, il Governo è intervenuto con prontezza e determinazione per creare uno stato di maggiore serenità nel Paese e, in particolare, per le imprese, i singoli cittadini e i vari investitori.

In questo senso considerato il notevole grado di integrazione dell'economia di tutti gli Stati membri che condividono un mercato unico e molte politiche comuni, una qualsiasi risposta alla crisi deve combinare gli aspetti monetari e creditizi,

la Lega Nord, attenta ai consumatori e alle piccole e medie imprese, aveva presentato degli emendamenti che andavano nel senso della limitazione all'erogazione del credito al consumo alle società di mediazione creditizia; creditizia; dei provvedimenti che andavano a introdurre sanzioni, anche penali, in caso di utilizzo di documentazione falsa da parte dei mediatori creditizi;

condividiamo quanto è stato previsto per garantire la liquidità del sistema e la continuità nell'erogazione del credito alle

il decreto al nostro esame è uno strumento per affrontare un aspetto specifico della crisi economica che stiamo conoscendo; questo questo aspetto specifico è dato dalla drammatica situazione di difficoltà nella quale versa il mercato finanziario e il vero e proprio rischio di collasso del sistema del credito connesso alle difficoltà del sistema finanziario. Un rischio di collasso, vorrei ricordare ai colleghi che hanno detto si tratta di un decreto necessario ma di fronte ad un rischio che è sostanzialmente già alle nostre spalle, che purtroppo non è alle nostre spalle. Nella capitale dell'economia globale, gli Stati Uniti d'America, penso si stia per manifestare un nuovo *tsunami* finanziario rappresentato dall'esplosione del tema delle carte di credito: ancora non abbiamo visto l'effetto potenzialmente devastante ed altrettanto pesante di quello determinatosi due mesi fa della esplosione di questo bubbone. Non ho intenzione in questo intervento di uscire da questo specifico, cioè la crisi dal lato della finanza, il sistema del credito, come affrontare i problemi che a questo proposito si propongono. Voglio però prima precisare un aspetto che viene troppo sottovalutato e che mi è sembrato sottovalutato anche nella discussione che si è svolta fin qui. Noi non abbiamo di fronte una crisi finanziaria che nasce nella finanza e che forse - come dicono alcuni - potrebbe trasmettersi all'economia reale come potrebbe non trasmettersi: il Presidente Presidente del Consiglio, per esempio, circa venti giorni fa, ha rassicurato gli italiani dicendo che non si trasmetterà. L'ha detto lui. La verità è che la crisi che abbiamo di fronte è una crisi economica che ha manifestazioni finanziarie; anzi, si è manifestata con effetti particolarmente devastanti sul versante finanziario, ma trova le sue ragioni di fondo nei grandi squilibri dell'economia globale.

e drammatica carenza di risparmio, che è stata alimentata da una costruzione dello sviluppo economico fondata sull'economia a debito; in particolare su un'economia a debito alimentata dai consumi delle famiglie, in un contesto nel quale la politica monetaria di intonazione enormemente espansiva delle autorità monetarie negli Stati Uniti d'America non ha fatto che alimentare questo bubbone. Di solito, succede che quando si determina una situazione di questo tipo si alzano i prezzi

e ha fatto da surrogato all'aumento dei prezzi, cioè all'inflazione generale - una gigantesca bolla immobiliare; senza questa naturalmente il sistema sarebbe esploso prima, con la bolla immobiliare ha tenuto più a lungo. un accenno di aumento del costo del denaro e lo sgonfiarsi della bolla speculativa sugli immobili hanno fatto venir meno nell'immediato alcuni capisaldi di questa economia del debito

carenza drammatica di risparmi: i deficit gemelli degli Stati Uniti. Poi si sente dire in giro che nessuno l'aveva previsto. Ma com'è possibile dire una cosa simile? Sono state scritte biblioteche sui deficit gemelli degli Stati Uniti: quelli delle famiglie quelli del sistema economico nel suo complesso dal punto di vista commerciale rispetto al resto del mondo. Lì si sono determinate le condizioni per l'esplosione della crisi. Dall'altro lato, in Asia, ma in particolare in Cina, si è registrata un'enorme eccedenza di risparmio:

La Cina è l'unico grande Paese in situazione di pace che abbia un livello di consumi delle famiglie inferiore al 40 per cento del prodotto interno lordo; attraverso questa strada persegue, con i *surplus* che si sono creati, disegni geostrategici che non hanno consentito che il *surplus* di risparmio della Cina si incontrasse, attraverso la politica monetaria ben condotta, con la carenza di risparmio degli Stati Uniti. Carenze di governo globale su questo versante, più scelte di politica economica e monetaria dei due Paesi hanno determinato le condizioni per l'esplosione

non si è rivelata una scelta particolarmente azzeccata, perché si è dato quell'esempio e tutti hanno pensato di poter essere potenzialmente coinvolti dallo stesso processo.

i pagamenti tra le imprese, tra i soggetti privati. Se non circola credito interbancario, molto banalmente, l'economia reale si ferma, non quella finanziaria come si sente raccontare. Il credito interbancario consente di far funzionare i pagamenti senza ricorrere al contante e senza ricorrere al baratto, signora Presidente, perché le uniche due alternative alla circolazione del credito tra le banche per consentire i pagamenti sono gli assegni o qualcosa di gli assegni o qualcosa di simile che consenta il pagamento non ricorrendo al contante, oppure il ricorso al baratto, non c'è un altro modo. Evidentemente, restituire fiducia nelle banche e quindi riavviare il credito interbancario era assolutamente indispensabile;

svolge una funzione cruciale nel sistema dei pagamenti, e quindi nel funzionamento del sistema economico di mercato, come le banche. O c'è credito interbancario o non c'è sistema economico funzionante, quindi non è vero che sarebbe sbagliato intervenire sulle banche perché poi si dovrebbe farlo anche in altri settori. Tutti i settori sono meritevoli di attenzione, ma è del tutto evidente che esiste un ruolo strategico del sistema finanziario per la ragione che ho detto.

a questa domanda è sì e no. Sì, perché una garanzia di ultima istanza da parte dello Stato per riavviare il sistema del credito interbancario, a mia conoscenza

perché la garanzia alle banche, fondamentale per riavviare il credito interbancario, come ho già detto, è funzionale a garantire alle imprese il flusso costante del credito di cui hanno bisogno per operare:

perché questo è funzionale; se le banche non ci fossero più, se fallissero, verrebbe meno lo strumento fondamentale per alimentare il processo produttivo. Tuttavia,

l'intervento a favore delle banche serva a riavviare il credito interbancario, in modo che il flusso del credito verso le imprese non si interrompa, non bisogna intervenire sulle banche, ma sulle garanzie a favore del credito delle aziende. Questo è chiarissimo; non c'è il minimo dubbio.

Altrove non hanno questo problema perché hanno un sistema basato su medie e grandi imprese; in Italia, invece, noi abbiamo - può piacere, a me piace, ad altri piace di meno - la piccola

facciamolo! La capacità di garantire dei consorzi fidi deve essere immediatamente triplicata, come minimo, attraverso un fondo specifico. Questa volta in bilancio bisogna prevedere una cifra

così. Rappresentante del Governo, la mia previsione è molto semplice. Si andrà verso una stagione nella quale ci sarà poco credito in giro a costi alti, oltre ad un enorme debito pubblico in giro per il mondo che cercherà risparmiatori disposti a comprarlo a condizioni vantaggiose, perché il debito pubblico aumenterà. In queste condizioni, il rischio che alle nostre imprese non arrivino i soldi necessari per il loro funzionamento è elevatissimo. Vi volete decidere o no a dar vita a questo fondo, a scriverlo in bilancio e almeno a

È questo lo spirito informatore che mi sembra si possa ravvisare nelle misure predisposte dal ministro Tremonti. E l'instabilità e variabilità della situazione finanziaria ed economica è dimostrata da vari indicatori. Oggi, ad esempio, le borse asiatiche sono calate del 6 per cento, il che vuol dire che non sappiamo domani cosa possa accadere alle borse europee e a Wall Street. C'è, quindi, una concatenazione tra un avvenimento e l'altro, difficilmente prevedibile e governabile. Pensiamo al prezzo del petrolio. Quando il prezzo saliva vertiginosamente tutti si auguravano che tornasse ai 50-60 dollari attuali. Ma mentre invece oggi ci si può rallegrare del diminuito prezzo del petrolio, considerata la costante interconnessione degli avvenimenti economici e finanziari, forse dobbiamo concludere che sarebbe stato preferibile un prezzo più alto e una crisi finanziaria in meno. meno. Il decreto-legge in esame fornisce il quadro normativo necessario per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione di misure straordinarie che dovessero rendersi necessarie, a causa delle ripercussioni legate all'attuale crisi finanziaria, per garantire la stabilità del sistema e e la tutela del risparmio. Tutto ciò nel rispetto dell'articolo 47 della Costituzione, del quadro di riferimento normativo nazionale, delle conclusioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea e dei successivi incontri internazionali, tutti favorevoli all'adozione di ogni misura necessaria per rinforzare il sistema bancario e proteggere i risparmi in presenza di crisi finanziarie in atto. L'intervento pubblico è effettuato solo in presenza delle esigenze di salvaguardia della stabilità e con la finalità di superare la situazione di difficoltà della banca ricapitalizzata. Le disposizioni recate dal provvedimento devono essere inquadrate nella prospettiva di una situazione finanziaria in grande evoluzione: infatti, a distanza di poche settimane dall'emergenza che ha dato origine al decreto-legge, risulta maggiormente evidente l'intento apprezzabile e condiviso attraverso il rafforzamento del sistema bancario di mettere in atto una serie di strumenti, anche innovativi e coraggiosi, per dare stabilità all'intero sistema e ridare fiducia ai risparmiatori e ai depositanti. Vero è che aver messo in campo, già a luglio scorso, da parte del Governo una manovra di consolidamento pluriennale dei conti pubblici, in grado di delineare un percorso credibile di controllo e di riduzione della spesa pubblica, ha fatto sì che l'Italia recuperasse credibilità sulla scena internazionale. Il provvedimento interviene con intelligenza su questioni di estrema delicatezza, quali l'intervento pubblico nel capitale delle banche ovvero la predisposizione di garanzie pubbliche per rafforzare i *ratio* patrimoniali e incrementarne la liquidità. Si tratta di misure che precostituiscono le basi per i prossimi provvedimenti volti a scongiurare una traslazione della crisi finanziaria sull'economia reale e la conseguente penalizzazione delle imprese. Quello che caratterizza in modo rilevante la misura predisposta dal Governo è la finalità primaria di salvare l'economia reale da una tempesta finanziaria frutto di una crisi di una finanza non creativa, ma artificiosa e nociva; tutto ciò attraverso misure serie e concrete. Le misure proposte dal Governo, dunque, hanno anzitutto l'obiettivo di tutelare il risparmio e di rassicurare i depositanti e non certo quello di difendere i singoli banchieri o gli speculatori finanziari con un impianto che salvaguarda un bene costituzionalmente tutelato - il risparmio -, in un rapporto corretto e trasparente tra il mondo della politica e il sistema bancario. Rilevo che, nel ripristinare un equilibrio reale della finanza, non si vogliono penalizzare le banche in quanto tali, ma piuttosto ridimensionare il comportamento di alcuni banchieri più interessati al salvataggio delle *stock option* e di altri prodotti simili.

e la mancanza di misure mirate a cambiare direzione ha portato agli eventi drammatici degli ultimi giorni e mesi. Le autorità si trovano ora a correre da un fuoco all'altro, mentre diventa sempre più evidente che il buco creato dalla speculazione non può essere colmato in un breve lasso di tempo. allora il tempo di cambiare rotta. Come ha più volte avuto modo di sottolineare il ministro Tremonti, oggi, lontani mille miglia dai giganteschi conflitti d'interesse di istituti bancari cresciuti a dismisura nel mondo globalizzato, nel nostro Paese noi dobbiamo capire insieme che siamo stati posti all'improvviso di fronte al bivio di una scelta economico-finanziaria che non consente esitazioni. Le banche d'affari hanno troppo spesso saputo generare ricchezza che poi è risultata illusoria. Anche in una fase indubbiamente difficile dell'economia italiana il Governo agisce, con il *placet* delle organizzazioni internazionali, con l'obiettivo di dare ossigeno ai mercati e di intervenire sull'economia per garantire una ripresa della produzione e per evitare lo spettro della recessione. Naturalmente - torno a ripetere - tutto ciò può compiersi perché il Governo ha effettuato un intervento importante di politica economica prima dell'estate con la manovra triennale: ha messo al sicuro i conti e si è garantito una credibilità internazionale che lo mette oggi in condizione di rappresentare l'Italia nei consessi internazionali dichiarando che abbiamo fatto quello che dovevamo e che siamo oggi pronti ad affrontare la crisi che si presenta nel nostro Paese. Paese. Non dobbiamo infatti dimenticare che siamo il Paese con il terzo debito del mondo, ma non siamo la terza potenza economica del mondo. Dobbiamo quindi affrontare le vicende della ripresa dell'economia nel nostro Paese tenendo presente l'enorme carico del debito pubblico, che costa alle casse dello Stato circa 75 miliardi di euro l'anno. Il Governo ha quindi operato questo intervento, che va visto nell'ambito di un ampio programma: prima la manovra di luglio, seguita dalla finanziaria al nostro esame, poi il disegno di legge sul federalismo fiscale e, infine, il disegno di legge anticrisi, presentato venerdì scorso nell'ultimo Consiglio dei ministri, a salvaguardia di famiglie e imprese. Voglio concludere con due riflessioni. Quanto alla prima, mi auguro che si tenga conto, in questo o in un altro provvedimento, di un sistema premiale, volto cioè a premiare le banche che hanno investito poco in titoli tossici, così da agevolare chi non ha speculato. Quanto alla seconda, intendo sottolineare con soddisfazione il fatto del provvedimento presso la Camera dei deputati, è stato soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 5, dove si prevedeva che, fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia, alle banche partecipate non si dovessero applicare le disposizioni speciali in materia di esercizio È rimasto quindi fermo il principio del cosiddetto voto capitario, che rappresenta un irrinunciabile presidio a tutela della specifica funzione esercitata dalle banche popolari. La crescita e la solidità creditizia delle banche popolari, infatti, sono oggi la vera garanzia di iniziative economiche valide, soprattutto delle piccole e medie imprese, che, in questa difficile congiuntura, possono assicurare la ripresa dello sviluppo del sistema Italia; laddove sono in crescita le banche popolari e di credito cooperativo, si registra un decremento delle grandi banche.

principalmente di restituire valore all'economia reale e a quelle categorie sociali che sono le vere protagoniste dello sviluppo del nostro Paese.

una proprietà che è di Telecom - società che a noi chiede, ad esempio, l'aumento del canone e che gode di un vantaggio forte, anche a detta dell'Unione europea, rispetto ad un servizio universale - non possa prendere in considerazione proposte costruttive.

di *news* e informazioni fuori dal suo gruppo (e non è comprensibile un fatto del genere), basterebbe rescindere il contratto di 6 milioni di euro con il canale CFN